onorevoli membri del Governo, cari colleghi, oggi parliamo dell'insufficienza venosa cronica cerebro-spinale, la ormai famosa CCSVI,

Questa sensazione, se all'inizio - come avviene spesso in ambito sanitario - poteva essere avvertita come un effetto placebo, ormai a distanza di anni e mantenendosi inalterata, diventa un fatto davvero positivo e, solo questo, giustifica un ottimo intervento. A questo si aggiunge il fatto che in questi anni

Signora Presidente, come i senatori interroganti sanno, il Ministero della salute segue con molta attenzione la questione delineata nell'interrogazione segnala che il Consiglio superiore di sanità (CSS), la più alta autorità sanitaria nel nostro Paese, ha affrontato le tematiche relative alla insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (CCSVI) e quindi alla «Nuova terapia endovascolare per la sclerosi multipla». Il CSS ha approfondito tale problematica, che ha destato l'interesse del mondo scientifico, nonché di numerose associazioni rappresentative dei malati di sclerosi multipla, ed ha così operato: ha costituito un gruppo di lavoro *ad hoc*; ha audito il professor Zamboni; ha espresso parere nella seduta dell'8 giugno 2010 ritenendo, all'unanimità, che «ad oggi l'efficacia di qualsiasi procedura terapeutica vascolare non è sicuramente dimostrata ed è quindi da posporre all'acquisizione di dati scientifici che provino una sicura associazione

Inoltre, il CSS nello stesso parere riteneva necessario «attendere i risultati di altri studi e in particolare di studi che, attraverso un approccio multimodale, dimostrino che la CCSVI è un'anomalia significativamente più frequente nella popolazione con SM rispetto ai soggetti di controllo. Qualora i risultati scientifici che emergeranno da tali studi dovessero dimostrare una sicura associazione epidemiologica e fisiopatologica tra la CCSVI e la sclerosi multipla,

di sanità ha ritenuto, sulla base dell'esame della letteratura scientifica, che, nonostante sia stata rilevata un'elevata associazione fra CCSVI e sclerosi multipla, non ne sia stato ancora dimostrato il nesso. Vanno pertanto perseguite sperimentazioni terapeutiche miranti a dimostrare che la riduzione o l'eliminazione della CCSVI porti a modifica della storia naturale della sclerosi multipla. Tale parere è altresì completato dalle seguenti considerazioni: «Le osservazioni preliminari di Zamboni e collaboratori sono di indubbio interesse e meritevoli di approfondimento con tutti gli strumenti che la ricerca medica ha oggi a disposizione e che, ai fini di una più adeguata valutazione dell'ipotesi medica in parola, devono essere resi disponibili: un *consensus* sulla metodica ultrasonografica da utilizzare per la valutazione del sistema venoso; un *panel* di esperti nel settore della diagnostica neurovascolare per fornire indicazioni riguardo all'esecuzione dell'esame e sui parametri da analizzare; uno studio in doppio cieco su soggetti normali di controllo, su soggetti asintomatici, ma con alterazioni ossee a livello della colonna cervicale, in pazienti neurologici affetti da sclerosi multipla e da altre patologie come l'amnesia globale transitoria, l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica, per valutare l'eventuale impatto della CCSVI su ogni patologia; la messa a punto di un protocollo diagnostico con un'ulteriore metodica di neuro-immagini convenzionali». Inoltre, considerato che: «la casistica studiata del professor Zamboni e presentata a supporto della sua ipotesi di forte correlazione tra CCSVI e risulta mancante di dati di riproducibilità della metodica, di dati sulla prevalenza della CCSVI in persone con sindrome clinicamente isolata o con forme di sclerosi multipla pediatrica che permettano di affermare che la CCSVI è presente nei pazienti che sviluppano dati ancora più recenti ottenuti da gruppi diversi da quello del professor Zamboni e presentati a convegni internazionali sembrano ridimensionare l'associazione tra CCSVI e la il Consiglio superiore di sanità ha quindi sottolineato che, per porre diagnosi di CCSVI, sono richiesti criteri definiti e condivisi dalla comunità scientifica. In particolare occorre, e cito nuovamente: «verificare mediante un approccio multimodale (risonanza magnetica ed ecodoppler) la presenza della CCSVI in pazienti con sclerosi multipla di differente tipologia: forme con sindrome clinicamente isolata (CIS), forme recidivanti-remittenti (RR), forme secondariamente progressive (SP), forme primariamente progressive (PP) e forme pediatriche; cronica) con la presenza di depositi di ferro, indagata mediante metodiche avanzate di RMN (risonanza magnetica nucleare); mettere in relazione i dati strumentali con gli aspetti clinici ed il decorso della malattia per valutare il ruolo eziopatogenetico del fenomeno». Il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto importante che qualificati gruppi di ricerca clinica interessati a queste problematiche pianifichino studi metodologicamente ineccepibili,

Infine, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato che, ed anche qui cito: «è stata anche proposta una nuova terapia del trattamento della sclerosi multipla che consisterebbe in una angioplastica endovascolare con palloncino; l'inserimento di uno *stent* è stato suggerito come "logica alternativa" per l'alto tasso di re-stenosi; tale procedura è stata già eseguita su un ridotto numero di pazienti con esito fatale in due casi; la piccola dimensione del campione, la mancanza di controlli, le *unblinded*-valutazioni neurologiche, il significativo processo di re-stenosi e inconsistenti protocolli della risonanza magnetica limitano l'interpretazione dei dati; ogni interpretazione sull'efficacia è resa ancora più debole poiché tutti i pazienti hanno proseguito immodificate le terapie originali; lo stesso professor Zamboni ha dichiarato che il trattamento endovascolare della CCSVI nella sclerosi multipla è ancora prematuro». Il Consiglio superiore di sanità si è riunito il 13 luglio 2010 per ascoltare in audizione le delegazioni delle principali associazioni di malati di sclerosi multipla. In tale sede è stata, in particolare, sollecitata una riflessione sulla possibilità che, indipendentemente da una presunta correlazione con la la CCSVI sia riconosciuta quale patologia-autonoma anche in Italia, con conseguente sottoposizione ad intervento di coloro i quali ne siano affetti. Il 19 gennaio 2011 il Consiglio superiore di sanità ha convocato in audizione le società scientifiche competenti, al fine di acquisire utili elementi per il prosieguo del dibattito così riaperto. Dalle audizioni sono emersi i seguenti elementi: cronica), descritta dal professor Zamboni, sarebbe diagnosticabile con indagini ultrasonografiche in base ai criteri pubblicati, che prevedono la positività di almeno due criteri sui cinque rilevabili; i suddetti criteri non sono stati validati verso un esame *gold standard*, anche perché la flebografia (possibile *gold standard*) è esame anch'esso soggetto a variabilità, in relazione alla pressione di introduzione del mezzo di contrasto, alla posizione del paziente, ad altre variabili interindividuali e alle apparecchiature utilizzate; gli stessi criteri non sono stati validati circa il loro valore predittivo nei confronti di alterazioni dell'emodinamica cerebrale già note in letteratura; tra i cinque criteri previsti per la diagnosi di CCSVI, uno prevede l'utilizzo dell'ecografia transcranica, attraverso una finestra ossea (sopracondilare) mai utilizzata in letteratura e per la quale mancano dati metodologici; l'esistenza della CCSVI e le correlazioni etiopatogenetiche collegate alla stessa sono ancora controverse e, pertanto, risultano necessari ulteriori studi, condotti con strumentazione adeguata, rigorosa metodologia di indagine e corretta selezione dei pazienti. Il 25 febbraio 2011 il CSS ha espresso all'unanimità un ulteriore parere sulla insufficienza venosa cerebro-spinale cronica e sulla sclerosi multipla, specificando, fra l'altro, che nella nota del Ministro della salute del 27 ottobre 2010, inviata agli assessori regionali alla sanità, contenente gli elementi conoscitivi e valutativi su sclerosi multipla e CCSVI, formulati da un apposito gruppo di lavoro, la dizione «si segnala che l'attuale sistema sanitario garantisce, in regime ospedaliero, sotto la responsabilità del medico, l'erogazione di terapie atte a diagnosticare, monitorare e, se indicato, correggere terapeuticamente anomalie dell'apparato

cito - «che, ad oggi, la CCSVI non possa essere riconosciuta come entità nosologica; che, ad oggi, non sia dimostrata la sua correlazione epidemiologica con la sclerosi multipla e, pertanto, l'intervento di correzione vascolare non può essere indicato nei pazienti affetti da tale patologia; che sia necessaria, invece, un'indicazione clinica chiara e netta, indipendentemente dalla presenza o meno di sclerosi multipla, per l'erogazione di misure atte a diagnosticare, monitorare e correggere anomalie dell'apparato vascolare venoso, qualora indicato, a causa di condizioni patologiche ad esse sicuramente riferibili». Nello stesso parere il CSS ha affermato la necessità che «eventuali procedure di correzione di patologia venosa in pazienti con sclerosi multipla siano effettuate solo ed esclusivamente nell'ambito di studi clinici controllati e randomizzati, approvati da comitati etici,

gli *end point* primari e secondari, il monitoraggio degli eventi avversi, le modalità e la cadenza del *follow up* ed infine le caratteristiche dell'analisi statistica». Da ultimo, il CSS ha indicato l'opportunità che «sia contrastata ogni finalità puramente speculativa ed economica; debba essere fatto tutto il possibile per proteggere i pazienti da facili entusiasmi, da speculazioni economiche e dai rischi connessi al trattamento stesso, ricordando che la ricerca biomedica e la pratica clinica devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità psicofisica della persona». Il parere di cui abbiamo letto ampi stralci è stato trasmesso, con nota a firma del Ministro della salute, professor Fazio, in data 4 marzo 2001, a tutti gli assessori regionali alla sanità, affinché se ne tenga conto nella predisposizione delle connesse attività di studio e assistenza e ai fini di una appropriata divulgazione. Mi sembra evidente che non sia il caso di parlare

per la lettura della cronistoria di quello che è successo al Consiglio superiore di sanità. Forse dal Ministero, in questo caso rappresentato dal Sottosegretario, mi sarei aspettata qualcosa di più, da un punto di vista politico. Ovviamente non siamo qui a validare studi scientifici e tanto meno a sostenere se quella sia la cura per una patologia piuttosto che un'altra; questo è compito ovviamente

Parliamo di numeri importanti. Nel mondo sono circa 1,3 milioni i pazienti: in Europa 400.000, in Italia 58.000, e di questi 22.000 circa potrebbero ottenere giovamento da quel tipo di intervento. Si parla di interessi, e credo che anche questo sia bene prenderlo in considerazione. Un malato costa, in farmaci, circa 80.000 euro all'anno.

ci ha descritto la sua ricerca come una ricerca *non profit*, che «si scontra con un interesse, un mercato che nei Paesi cosiddetti progrediti è di un miliardo di euro al mese. Capirete che ritardare di un mese rende un miliardo e, quindi, va bene. Tuttavia, proprio per la responsabilità che dobbiamo avere nei confronti dei cittadini e dei pazienti, è inaccettabile che la ricerca possa essere ostacolata, o fuorviata, da dati rilevati in un modo non rigoroso». Io credo che, innanzitutto, da un punto di vista politico dovremmo chiederci quale tipo di studi stiamo portando avanti in Italia e in che tipo di centri stiamo inviando i pazienti;

chi ne ha la possibilità. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, e vanno dalla fecondazione assistita, alla conservazione del cordone ombelicale, alla RU486, alla ricerca con le cellule staminali ed embrionali, all'eutanasia e al testamento biologico. Quindi, per quanto mi riguarda, io non mi ritengo soddisfatta della risposta, anche perché

qui presente di essere una persona che ha sempre dimostrato grande sensibilità, e su questo vorrei soffermarmi.

la CCSVI coincida con la sclerosi multipla; ha solo rilevato dei miglioramenti che chiunque di noi, se conosce dei pazienti che si sono sottoposti a questo

quelli che, sempre sotto il controllo dei comitati etici, stanno procedendo, di fatto anche vietando alle università

di mezzi, metodi e numeri nettamente superiori, si approprieranno di un qualcosa che è cresciuto in Italia, che può esaltare la scienza italiana, che chiede semplicemente di intervenire su tale patologia.

Il fenomeno legato al commercio dei medicinali contraffatti non può essere ridotto a una mera questione numerica, in quanto si tratta di un fenomeno sotterraneo e spesso legato alle attività della criminalità organizzata. I dati in possesso dell'AIFA sono da considerarsi meramente indicativi. Nonostante ciò, faccio presente che, secondo stime ufficiose, la percentuale di farmaci contraffati in Europa sarebbe pari all'1 per cento, mentre in Italia l'incidenza di tale mercato sarebbe di dieci volte inferiore anche grazie alla rete di distribuzione italiana e al divieto della vendita *on line*. La comunicazione al pubblico, relativamente ai rischi legati all'acquisto di farmaci attraverso Internet, costituisce una delle fondamentali iniziative di contrasto al fenomeno della contraffazione. di ottobre 2009 il Ministero della salute, in collaborazione con l'AIFA, l'Istituto superiore di sanità e le altre istituzioni che fanno parte della *task force* anticontraffazione Impact Italia, hanno ideato e realizzato una campagna di sensibilizzazione durante la quale sono stati distribuiti in circa 75.000 farmacie degli opuscoli contenenti informazioni sui rischi legati all'acquisto di medicinali mediante farmacie *on line* illegali. In particolare, gli obiettivi della campagna di comunicazione sono stati i seguenti: informare sui rischi per la salute; scoraggiare il paziente ad acquistare i farmaci tramite le farmacie *on line* o presso canali non autorizzati non autorizzati (come palestre, *sexy shop* o centri estetici); supportare e divulgare il messaggio che i farmaci acquistati in farmacia e negli esercizi commerciali nei quali è concessa la vendita di farmaci da banco e di automedicazione non possono essere contraffatti; fornire al paziente informazioni minime di valutazione del rischio (quali la presenza del bollino ottico su tutte le confezioni di farmaci autorizzati in Italia e la possibilità di verificare la tracciabilità, se l'acquisto del farmaco stia avvenendo da un soggetto autorizzato alla vendita di farmaci al pubblico; indirizzare il paziente, in caso di sospetto e incauto acquisto di un farmaco contraffatto, invitandolo a collegarsi al sito Impact Italia. Nell'ambito della campagna di comunicazione, è stato inoltre realizzato dall'Istituto superiore di sanità il sito governativo di Impact Italia (www.impactitalia.gov.it). Il sito rappresenta un importante strumento di collegamento tra autorità e cittadino. I principali obiettivi sono, infatti, quelli di informare il cittadino sulla reale entità e diffusione della contraffazione farmaceutica e sui rischi derivanti dall'assunzione di farmaci contraffatti, di scoraggiarlo dall'acquistare farmaci tramite le farmacie *on line* o da altri canali non autorizzati e, allo stesso tempo, di renderlo compartecipe alle azioni di contrasto all'ingresso e alla circolazione di farmaci contraffatti in Italia. Per questo scopo sono stati appositamente ideati due sportelli *on line* aperti al pubblico: uno per segnalare a Impact Italia casi, anche solo sospetti, di farmaci contraffatti con i quali il cittadino possa essere entrato in contatto, l'altro per porre quesiti specifici sul problema della contraffazione farmaceutica. Le segnalazioni relative al rinvenimento di un farmaco contraffatto e le domande dei cittadini sul tema della contraffazione farmaceutica sono gestite attraverso un *network* collaborativo che consente l'interconnessione delle istituzioni governative che partecipano alle attività di Impact Italia e la loro cooperazione *on line* attraverso lo scambio in tempo reale di comunicazioni, informazioni e documenti. Sono attualmente in fase di sviluppo campagne *web* indirizzate a *target* specifici. Alla luce dei positivi risultati ottenuti in termini di sensibilizzazione del pubblico, sono in via di realizzazione altre iniziative simili, come la campagna di comunicazione rivolta ai più giovani, che nel nostro Paese rappresentano larga parte degli internauti e che sono più esposti al pericolo delle farmacie *on line* illegali. Nella consapevolezza che una corretta informazione in questo campo è fondamentale e indispensabile per scoraggiare forme di automedicazione che potrebbero alimentare il fenomeno della vendita di farmaci su Internet, l'AIFA nel settembre 2010 ha realizzato, in collaborazione con un ente di ricerca, una indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana volta a tracciare un quadro reale degli atteggiamenti e comportamenti degli italiani rispetto agli acquisti *on line* di farmaci. I risultati ottenuti verranno utilizzati per definire un'ulteriore campagna volta a scoraggiare queste forme di acquisto e a promuovere, altresì, il ricorso adeguato e consapevole ai medicinali. Peraltro, l'Agenzia ritiene che il fenomeno illegale della diffusione dei medicinali contraffatti incida principalmente sulla tutela della salute pubblica e che esso non potrebbe essere ridotto drasticamente agendo sui brevetti. Il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, interviene continuamente nel controllo e nella censura della pubblicità non corretta. Le iniziative di *intelligence* informatica realizzate dall'AIFA, unitamente al Ministero della salute e alle altre istituzioni interessate, l'impegno profuso a livello nazionale e internazionale per inserire norme più severe dal punto di vista della prevenzione e del contrasto (come la recente operazione anticontraffazione «Pangea III») hanno consentito di intervenire direttamente e chiudere alcune farmacie *on line* illegali.

nel campo della sanità, che veda in primo piano coinvolti l'organizzazione territoriale, le direzioni nazionale e regionale del Servizio sanitario e il sistema delle farmacie. Abbiamo bisogno di fare una informazione molto più capillare, che porti a contatto con tutte le persone, specialmente le più fragili e deboli, affinché possano verificare il loro investimento su farmaci di dubbia o di semplificata utilità nell'immediatezza della risposta che possono dare ai bisogni. Mettere in guardia l'opinione pubblica rispetto a questo, mi sembra un dovere permanente. Concludo dicendo che noi, in questo momento, sappiamo che abbiamo a che fare con un impianto complessivo della nostra società. Se colleghiamo gli interessi di mercato gli interessi pubblicitari, tra loro molto connessi (e quindi spesso pubblicità disonesta),

diversi da quelli della salute, dei farmaci, notiamo che c'è un crogiolo di interessi che sono esattamente il contrario di quello che ci ricorda sempre la Costituzione con il suo articolo 32. Abbiamo quindi il dovere di essere molto più competenti competenti e diffusi negli interventi di conoscenza e di informazione di quanto non siamo allo stato attuale. Comunque, ringrazio

come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» stabilisce che l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia. L'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» prevede, al comma 1-*bis*, che l'indennizzo di cui all'articolo 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme succitate, nelle forme succitate, nati negli anni dal 1959 al 1965. Il decreto n. 163 del 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante il regolamento dì esecuzione delle legge n. 244 del 2007, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide,

presentino le relative domande al Ministero, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007. La documentazione sanitaria da allegare alla domanda è indicata nelle linee guida per l'istruttoria delle domande, emanate con circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 5 novembre 2009, n. 31. Le domande, corredate della documentazione di cui al regolamento e alla circolare, vengono trasmesse da questo Ministero alle commissioni mediche ospedaliere affinché esprimano il giudizio sanitario procedendo secondo modalità operative analoghe a quelle stabilite per l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992. In data 19 maggio 2010 il Ministero inviava una nota all'Istituto superiore di sanità, con la quale si evidenziava che, dall'esame dei verbali pervenuti dalle commissioni competenti a esprimere il giudizio sanitario, era emersa una importante difformità tra gli stessi, relativamente ai criteri di valutazione seguiti. In taluni casi, si valuta il giudizio non esprimibile, in quanto condizionato alla presentazione di una documentazione che ormai, a più di quarant'anni di distanza dall'evento, non è reperibile. L'Istituto veniva invitato a fornire elementi informativi, al fine di supportare con utili strumenti di valutazione l'attività delle commissioni e ad esprimersi sull'eventualità di apportare correttivi alla normativa di settore. L'Istituto superiore di sanità trasmetteva al Ministero il parere richiesto il 1° luglio 2010. 23 luglio si riuniva quindi il gruppo tecnico che aveva definito le linee guida applicative, recepite nella citata circolare 5 novembre 2009, n. 31. Il gruppo, preso atto della problematica relativa al giudizio sul nesso di causalità, che è stato valutato in numerosi casi non esprimibile, e acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, ha approvato un documento che individua un criterio tramite il quale si può evincere comunque la sussistenza del nesso causale. In data 29 luglio 2010, il Ministero della salute indirizzava al Ministero della difesa (da cui dipendono le commissioni competenti) una nota con le conclusioni del gruppo tecnico, invitando la direzione generale della sanità militare a dare indicazioni alle commissioni di tenerne conto nell'espressione del giudizio del nesso causale tra l'assunzione della talidomide da parte della madre e l'infermità. L'Amministrazione ha dovuto trovare la soluzione al problema della dimostrazione del nesso causale in un'ipotesi come quella della talidomide, che è descritta dalla dottrina come il tipico caso "di scuola", nel quale l'individuazione di una responsabilità di tipo risarcitorio risulta impossibile. Nell'esperienza in corso, di attuazione di un rimedio di tipo indennitario, si è palesata la necessità di contemperare due contrapposte esigenze: da un lato, quella di rendere effettivo il diritto all'indennizzo per tutti i soggetti che ne siano astrattamente titolari e, dall'altro, quella di evitare che anche soggetti affetti dalle patologie enumerate dalla legge, e tuttavia non causate dalla somministrazione del farmaco talidomide, possano beneficiare dell'indennizzo. Il tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la trasmissione della documentazione alle commissioni competenti è dovuto alla descritta necessità di approfondire ulteriormente il criterio tecnico-scientifico da utilizzare nella valutazione dell'esistenza del nesso causale, che nel caso in discussione non può soddisfare i criteri medico-legali classici, essendo trascorsi più di quarant'anni dalla commercializzazione del farmaco, con una difficoltà oggettiva da parte della maggioranza degli istanti a reperire la documentazione sanitaria attestante l'assunzione dello stesso farmaco durante la gestazione. se l'Amministrazione non avesse operato in tal senso, coinvolgendo l'Istituto superiore di sanità, il gruppo tecnico e il Ministero della difesa, una quota significativa di questi soggetti avrebbe visto preclusa la possibilità di accedere ai benefici spettanti. Per quanto riguarda gli aspetti della problematica in esame che riguardano specialità medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha inteso precisare che dal riscontro effettuato sulla rete, risulta che dei farmaci autorizzati contenenti talidomide, nel periodo indicato nell'interrogazione in esame, non vi è più traccia nei sistemi informatici dell'AIFA. L'Agenzia sottolinea che poter definire con precisione il periodo di effettiva commercializzazione in Italia dei farmaci a base di talidomide è oggi praticamente impossibile, in considerazione del fatto che, tra l'altro, le società interessate sono ormai scomparse o sono state incorporate da aziende più grandi. Peraltro, data l'estrema gravità della situazione, si può ritenere verosimile che, all'epoca, sia stato applicato l'articolo 28 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, che dava facoltà al Ministero dell'interno di proibire la vendita al pubblico e disporre il sequestro delle specialità medicinali revocate. Per quanto di interesse, si mette a disposizione dell'Assemblea un elenco delle specialità medicinali a base di talidomide che è stato possibile individuare.

è la prima volta che ringrazio un rappresentante del Governo per la risposta ad un'interrogazione parlamentare,

ma per la presenza in Aula del Governo su un tema che, a giudizio nostro e di molti, è stato ingiustamente sottovalutato nel nostro Paese.

2009) per il decreto ministeriale che ha poi definito il regolamento di attuazione con la connessa circolare esplicativa del Ministero.

riuniranno a Roma per fare tutti insieme il punto della situazione. Faccia in modo che il Governo riesca, per quella data, a mandare un messaggio di presenza, di tempestività e di ulteriore incisività di risposta.

mi riferisco all'interrogazione della senatrice Soliani in merito al crollo, avvenuto nella notte dell'8 dicembre 2010, di una parte del muro di cinta del Castello di Compiano,

il primo sopralluogo per accertare lo stato della compagine muraria a seguito del parziale crollo subito. Il tratto di cinta muraria del Castello crollato è, infatti, quello prospiciente prospiciente piazza della Cisterna ed interessa un fronte di metri 25 per una altezza media di metri 8. Particolarmente pericolanti ed a rischio di successivi crolli sono subito apparsi i tratti di cinta muraria che precedono e seguono la parte crollata ed interessano un fronte di 55 metri, sempre per una altezza di circa 8 metri. Nella stessa situazione appare inoltre la porzione di cinta muraria ad est per un tratto di circa 40-50 metri. I tecnici hanno ragione di ritenere che la causa del crollo sia dovuta all'insaccamento di una grande quantità di acqua visto che, nei tre mesi precedenti il crollo, il territorio del Comune di Compiano è stato interessato da piogge molto intense, gelate notturne e scioglimento repentino della neve a causa della pioggia battente. Durante il sopralluogo della soprintendenza è emerso che i primi presidi di messa in sicurezza delle cortine dissestate - ad eccezione di quelli a protezione del sottostante

che opererà gli interventi di puntellamento. Durante il sopralluogo non è stata consegnata alcuna iniziale valutazione sugli interventi di restauro della cortina muraria. È da evidenziare tuttavia - al fine delle valutazioni complessive sullo stato di conservazione che interessa l'importante ricetto definito, assieme al suo borgo antico, fra i più interessanti contesti castellani italiani - che ulteriori criticità sono state rilevate anche presso il torrione a nord del Castello, il quale presenta evidenti crepe verticali in sommità, proprio dove la muratura evidenzia chiare zone ove l'allettamento di malte è stato eroso dal tempo. Inoltre, è stato evidenziato che, già in occasione degli interventi di riqualificazione dell'area «Le Porte» (area di accesso principale al borgo) circa

di anni precedenti da destinare ad edifici non statali, come è appunto il Castello di Compiano. La esigua disponibilità dei fondi 2011, per il restauro di beni architettonici in generale e segnatamente per quelli non statali, non ne ha consentito, per il momento, l'inserimento nel piano ordinario di spesa dei lavori pubblici, attualmente in fase di adozione. I competenti uffici periferici del Ministero avevano peraltro assicurato la consulenza ed il supporto scientifico per ogni iniziativa di restauro con proventi derivanti da sponsorizzazioni o accordi con enti locali. In data 10 febbraio, infatti, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza ha effettuato un sopralluogo, unitamente al tecnico comunale e all'ingegnere del servizio tecnico di bacino di zona della Regione Emilia Romagna, per accertare l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza delle parti crollate e di quelle limitrofe. In quella stessa occasione si è appresa l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione per la progettazione dell'intervento relativo alla fase ricostruttiva del tratto murario crollato di circa 20 metri di sviluppo lineare, tra il Comune di Compiano e il servizio tecnico della Regione. Dallo stesso servizio tecnico si è altresì appreso che la Regione Emilia Romagna, per il tramite dell'Agenzia di protezione civile, ha già concesso due finanziamenti di 30.000 e 35.000 euro (su risorse rese disponibili dalla legge regionale n. 1 del 2005, articolo 10), per consentire la rimozione e la conservazione del materiale in pietra crollato in vista del suo riutilizzo.

nell'immediato, secondo una stima di massima, effettuata proprio dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza,

Da questo punto di vista credo che meriti una riflessione l'indicazione fornita dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna,

molto sottolineato - che non solo avete guardato e preso in mano la situazione, ma adesso la portate avanti e date anche il vostro contributo, perché senza il contributo del Ministero per i beni culturali le istituzioni locali da sole non ce

culturali*. Mi riferisco all'interrogazione del senatore Pedica con la quale si chiedono notizie in merito ad un'area in via Nomentana, in un tratto ricadente nei Municipi IV e V del Comune di Roma, nella quale egli riferisce sono stati costruiti abusivamente capannoni ad uso commerciale. Vorrei individuare, a tale riguardo, le aree interessate dall'interrogazione parlamentare. Area ricadente nel Municipio IV: la zona è soggetta a diversi dispositivi di tutela previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), parti II e III, sia sotto il profilo monumentale che paesaggistico, nonché a provvedimenti di tutela archeologica limitatamente al lotto corrispondente al n. civico 1125 di proprietà della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (Propaganda Fide). Nel tratto compreso fra i chilometri 10,600 e 11,300 numerosi capannoni ad uso commerciale sono sorti in violazione delle norme urbanistiche. Tuttavia, da un punto di vista archeologico, anche in caso di procedura regolare non si sarebbe potuto esprimere un parere di diniego a priori ma solo avanzare una richiesta una richiesta di saggi preventivi. In senso generale, tuttavia, la Soprintendenza archeologica di Roma ha più volte espresso giudizi negativi o quantomeno perplessità sull'uso degli spazi posto in essere nell'area. Parte delle strutture realizzate sia sul lato meridionale (di proprietà di Propaganda Fide) sia sull'opposto lato settentrionale, in cui la proprietà è suddivisa tra la Società agricola immobiliare Riserva della Cecchina e la la Propaganda Fide, sono riconducibili al nominativo Lucarelli, che ha tra l'altro eseguito scavi non autorizzati di posa cavi nella fascia densa di tombe prossima al tracciato della via Nomentana, per alcuni dei quali si attende ancora il completamento degli accertamenti imposti nel 2008. Area ricadente nel Municipio V: diversamente l'area interessata dalla demolizione, ubicata nel Municipio V, in corrispondenza di via Nomentana 1100, sempre di proprietà di Propaganda Fide, non è sottoposta a vincolo monumentale o paesaggistico ai sensi della II o della III parte del Codice dei beni culturali e paesaggistici. L'area non risulta sottoposta neanche a tutela archeologica in quanto la proposta di perimetrazione, *ex* articolo 142, 1, lettera *m)* (ovvero il vincolo paesaggistico su zone di interesse archeologico previsto dal Codice), denominata Fosso di San Basilio-Parco di Aguzzano e pubblicata il 19 dicembre 2002, è decaduta. Nondimeno, anche in assenza di vincoli, la zona è stata sempre monitorata dagli uffici presenti sul territorio, in particolare, relativamente al civico 1100, su segnalazione della Soprintendenza archeologica. Il Comando del V Gruppo dei vigili urbani ha constatato nel 1996 la realizzazione di una recinzione in assenza di prevista autorizzazione ed un aumento della superficie destinata ad esposizione a cielo aperto. Nel mese di novembre 2001, presso lo stesso civico, la società Centro risparmio srl - il cui legale rappresentate risulta essere Emiliano Lucarelli - ha realizzato una trincea per la messa in opera di una nuova recinzione la stessa Soprintendenza ha effettuato in due riprese - novembre 2001 e gennaio 2002 - delle indagini di verifica con esito negativo. Dalla documentazione relativa alla DIA trasmessa dalla società Centro risparmio si si apprende che per l'immobile di via Nomentana 1100-1102 è stata presentata domanda di sanatoria edilizia in data 31 dicembre 1986, ma agli atti della stessa Soprintendenza archeologica tale domanda non risulta trasmessa dall'Ufficio condono edilizio del Comune di Roma. Peraltro si rappresenta che non risultano agli atti segnalazioni di incendi nel territorio del Municipio V e va riferito che il programma di recupero urbano San Basilio, *ex* articolo 11 della legge n. 489 del 1993, prevedeva la demolizione degli insediamenti abusivi lungo i due lati della via Nomentana - per un totale di 53.000 metri cubi - ed il loro ricollocamento all'interno di un vasto edificio commerciale da realizzare a San Basilio. Anche la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma ha disposto un sopralluogo sull'area. È stata l'accertata inesistenza, allo stato attuale, di volumetrie sull'area anche se, da un riscontro effettuato sulla base di riprese aeree di *Google Earth*, i capannoni risultano esistenti nel volo effettuato in data 22 settembre 2006, mentre non sono più rappresentati in quello successivo del 29 luglio 2007. Si presume, pertanto, che la demolizione dei capannoni, di cui è rimasta traccia nel sedime di cemento, sia stata realizzata tra il settembre 2006 e il luglio 2007. Risulterebbe, infine, che parte delle attività sia stata spostata nel territorio del Municipio IV in edifici preesistenti, ma l'area è sottoposta a tutela non comprensiva dell'aspetto archeologico. Interventi anche recenti, relativi principalmente a opere pubbliche, hanno determinato nella fascia contigua alla via Nomentana ritrovamenti archeologici specialmente di tombe, puntualmente sottratte alla distruzione, anche con l'imposizione di varianti; alla tutela di fatto delle aree puntiformi faranno seguito i provvedimenti formali. Concludo sottolineando che, ogni qual volta le aree presentino un interesse in qualsiasi modo legato alla competenza di questo Ministero e, quindi, non ricadano sotto la sola competenza municipale, l'azione degli uffici territoriali sarà sempre opportuna e puntuale.

nota di risposta della Sovrintendenza archeologica di Roma, ossia dei funzionari che risultano competenti per il territorio, sia del IV che del V Municipio, per verificare se sussistano o meno i vincoli ambientali e archeologici, rispetto ai quali lei in parte mi ha risposto.

da accertamenti fatti presso i municipi di competenza e da indagini territoriali, che, proprio dove è presente il capannone del signor Lucarelli, persistono ancora oggi vincoli ambientali impeditivi al rilascio del condono edilizio. E questa

e anche al numero civico 1100 di via Nomentana, ancora oggi sussistono istanze di condono edilizio a sanatoria di fabbricati abusivi, depositate presso l'Ufficio del condono edilizio, nonostante gli stessi, come lei ha detto, siano stati rimossi già dal 2007.

la richiesta di condono ma non esistono i capannoni; c'è allora qualcosa che non riusciamo a capire. Un nesso comunque ci deve essere, ma non lo capiamo. Sicuramente qualcosa di speculativo c'è, ma ancora non è chiaro dalla sua risposta e non è quindi chiaro neanche quello che dovrò andare a fare da domani in poi. Sicuramente solleciterò lei, che è stato molto attento a rispondere a questa mia interrogazione, però bisogna che andiamo insieme sul luogo per verificare, magari anche interrogando direttamente il signor Lucarelli. Ripeto, leggendo le carte, mentre lei giustamente ci relazionava, mi mancano degli elementi per dire: «Grazie, signor Sottosegretario, è stato esaustivo». Abbiamo parlato di questo argomento e lei ha risposto, ma lo ha fatto sostanzialmente